Onorevole Presidente, La informo che il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data odierna, adottati su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Sandro BONDI dalla carica di Ministro per i beni e le attività culturali, ha nominato Ministro del medesimo Dicastero il dott. Giancarlo GALAN, il quale cessa dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ed ha infine nominato l'on. Dott. Francesco Saverio ROMANO Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. F. to Silvio Berlusconi» Ringrazio il sottosegretario Crosetto, che ci consente con la sua presenza di poter svolgere i nostri lavori

l'occasione della conversione in legge del decreto ha consentito un dibattito che, al di là della sottolineatura sul ritardo del provvedimento, sia in sede di emanazione sia in sede di conversione, ha dato l'opportunità ai Gruppi di una riflessione su quel che è accaduto, sul sentimento nazionale che si è manifestato il 17 marzo, sul confronto che si è aperto sul tema dell'Unità nazionale. Io credo sia opportuno recuperare alcune riflessioni, sia pur brevemente, a partire da una valutazione che in particolare mi ha colpito nel corso del dibattito, quella del rappresentante della Lega, il senatore Garavaglia, che ha posto una questione a mio avviso cruciale, cioè di come oggi si recupera una visione, una missione, una strategia, un'idea guida, un'idea forza che possa caratterizzare i 150 anni dell'Unità nazionale, consentendo di guardare alla prospettiva futura, a come cioè si realizza, dopo 150 anni, la modernizzazione istituzionale italiana intesa come una grande occasione per la ripresa del sistema Paese. Il senatore Garavaglia individuava questa idea forza, questa idea guida, questo motore della modernizzazione nel federalismo, nell'esigenza cioè di dar vita a questa grande riforma che peraltro è l'obiettivo storico di una forza politica.

Se io dovessi trovare un'ulteriore definizione alla riflessione del senatore Garavaglia, direi che oggi la sfida che abbiamo di fronte sul terreno istituzionale e sul terreno economico-sociale è quella di dar vita ad un nuovo grande patto patto nazionale, che rafforzi l'unità o, se si vuole, che realizzi l'unità, superando i disequilibri, le differenzee i deficit che ancora accompagnano la dualità del sistema Paese e, dentro questa dualità, l'esigenza di crescita del Mezzogiorno, nella consapevolezza che, se cresce il Sud, cresce l'Italia. Da questo punto di vista e per senso di responsabilità, il riferimento che il presidente della Repubblica Napolitano ha fatto nel suo pregevole intervento alla Camera dei deputati ci deve guidare esattamente lungo questa riflessione. Io di quella riflessione colgo la parte più critica a proposito del Mezzogiorno e dei meridionali: il fatto che, con la questione meridionale, debbono innanzitutto far conto e debbono innanzitutto trovare senso di responsabilità e capacità di qualità di classe dirigente i meridionali ed il Mezzogiorno, pur dentro un quadro di riferimento storico che certamente non ha aiutato il rapporto tra masse e Stato e che certamente non ha portato a compimento il processo di nazionalizzazione delle masse dentro la costruzione dello Stato unitario. Resta aperta questa ferita storica nel rapporto tra Mezzogiorno e Stato, che determina ancora oggi una serie di conseguenze, e proprio per questo rende, anche da questo punto di vista, più forte e più significativa l'esigenza di una modernizzazione istituzionale per aprire una nuova fase costituente in cui, da Nord a Sud, si possa partecipare alla costruzione della prospettiva nazionale dell'Italia del domani e dell'Italia del futuro. Dal punto di vista della necessità di rafforzare questo ragionamento,

Quando oggi si fa questo forte richiamo all'unità, bisogna tener conto dell'impatto che ha determinato su questa visione unitaria e, in particolare, sul ruolo e sulla funzione dello Stato nazionale la riforma del Titolo V e l'idea di fare una riforma che ha trasformato la gerarchia istituzionale in orizzontalità istituzionale attraverso l'articolo 114 della Costituzione novellata, che ha messo sullo stesso piano, nell'unità della Repubblica, il Comune come lo Stato nazionale. Oggi ci rendiamo conto di quanto sia stato velleitario immaginare questa scelta, che ha ridotto lo Stato nazionale e gli ha tolto ruolo, funzione e competenza, proprio oggi che torna in maniera prorompente l'esigenza di riflettere intorno al ruolo e alla funzione dello Stato nazionale, per assumere quelle grandi politiche necessarie, da Nord a Sud, per raggiungere quegli obiettivi di cambiamento e di modernizzazione. Da questo punto di vista, la riflessione sul 17 marzo ci deve portare a costruire un percorso che renda davvero utile quel che si è determinato: non solo l'occasionalità celebrativa, ma una capacità forte di rendersi finalmente conto che il Paese

che di questa missione nazionale dovrebbero fare la bandiera per recuperare ruolo, funzione e cambiamento e per non farsi irretire dalla quotidianità, che corre il rischio di bloccare l'azione di rilancio e di modernizzazione che il Governo ha promesso agli italiani e che non sempre riesce a realizzare, proprio perché ha perso questo senso, questa visione e questa funzione. inizio con una puntualizzazione non puntigliosa e molto breve sul nostro emendamento, che era stato adottato dalla Commissione a proposito della giornata dell'indipendenza e dell'indivisibilità del Paese è stato considerato estemporaneo. Era tutt'altro che estemporaneo, perché era stato depositato il 9 marzo scorso, quindi assai prima del successo popolare della festa del 17 marzo, e riportava alla lettera il contenuto di un disegno di legge da noi depositato già a febbraio. Era stato dichiarato ammissibile e privo di oneri, nonché collocato, non nel decreto-legge, ma nell'articolo unico del disegno di legge di conversione, secondo il Regolamento. Ricordo che l'Italia non era indipendente prima del 1861 e che il 17 marzo di quell'anno è stato possibile proprio grazie alla Seconda guerra d'indipendenza.

e celebra l'Unità d'Italia. La festività del 2 giugno, proposta in alternativa nella polemica inutile, non riguarda l'indivisibilità, ma la forma repubblicana, perché

in cui, nel 1861, si riunì il primo Parlamento nazionale, ma questo fa parte di un discorso che affidiamo al futuro. Per celebrare con un voto positivo questo provvedimento, voglio ricordare che forse non sarebbe inutile ogni tanto tornare alla memoria delle fonti, al modo con cui gli uomini hanno combattuto nel momento della lotta per la costruzione dell'unità e dell'indivisibilità dell'Italia. Voglio ricordare figure meravigliosamente irregolari che sono state trasformate dalla visione paludata della storiografia encomiastica e che, viste da vicino, svelano come le persone che si sono date da fare per l'Unità d'Italia avessero dei profili che oggi forse potrebbero risultare davvero curiosi. D'Azeglio, fin oltre i 30 anni, ha pensato di essere essenzialmente un pittore paesaggista.

poligrafo, scrittore e ha vissuto esule per lunghi anni in Svizzera perché non poteva fare una vita normale in Italia, nella sua Lombardia. ha dedicato uno scritto mirabile sui caratteri naturali e civili, in cui, lo ricordo di sfuggita, parla con espressione straordinaria della "nostra patria artificiale". Questa idea della nostra patria artificiale rappresenta la capacità e la laboriosità di mutamento dell'opera dell'uomo su un territorio inospitale, basato sul disordine idraulico, che l'uomo ha regimato, ha trasformato in praterie coltivabili, in pianure boscate, non di boschi naturali, ma di piantate di alberi che servivano alla cultura umana. Poi c'è anche il Sud, che ha dato un contributo fondamentale all'Unità d'Italia. Ricordo la figura di Settembrini, Settembrini, repubblicano, insegnante, un personaggio straordinario, che sapeva tradurre dal greco al latino e dal latino al greco senza passare dall'italiano.

Personaggi che non hanno nulla di costituito, di paludato; personaggi che hanno vissuto con difficoltà. Quando Cattaneo fu nominato senatore, poiché era un repubblicano, si rifiutò di giurare fedeltà al re e non partecipò mai alla vita senatoriale. quando si ricorda l'Unità d'Italia bisognerebbe ricordare anche le originalità che ne hanno costituito la potenza generatrice. Lo spirito del Risorgimento e della visione delle fonti ci dovrebbe ricordare con senso autocritico - poiché il senso dell'unità, dell'indipendenza e dell'indivisibilità del Paese si poggia anche sulla riflessione critica - anche i cannoni di Bava Beccaris

Eventi che sono stati ricordati da pagine che restano luminose nella nostra storia. Il simbolo della Prima guerra mondiale è «Un anno sull'altopiano» di Emilio Lussu: un eroe militare volontario in guerra che scopre durante la guerra che bisogna cambiare idea, che la guerra è una cosa orribile;

Insieme a lui, Nuto Revelli che, durante il ritorno dal Don, porta via un parabellum, un'arma russa eccezionale, con l'intenzione ferrea di servirsene nella riconquista della democrazia in Italia. Cosa che farà. È così, attraverso queste figure che si allacciano l'una all'altra, che lo spirito del Risorgimento si congiunge con lo spirito della Resistenza. Voglio concludere ricordando un verso che spesso è stato interpretato come manifestazione del moralismo manzoniano: «Il santo Vero mai non tradir: né proferir mai verbo, che plauda al vizio, o la virtù derida», un verso tutt'altro che moralistico che contiene in sé lo spirito dell'Illuminismo con cui Manzoni celebrava Carlo Imbonati. È una visione laica (non inganni l'aggettivo «santo») della verità e dei doveri civili. Quel verso chi volesse potrebbe facilmente connetterlo alla nobiltà dell'articolo 54 della Costituzione dove si dice che chi è incaricato di compito pubblico deve svolgere il suo compito con disciplina ed onore (cosa che il Capo di Governo sembra incapace di concepire). È in nome della nobiltà di queste idee e di questi ricordi che il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà a favore di questo provvedimento.

del mio Gruppo. Lo faccio con gioia e con grande fierezza. Lo faccio da italiano, da italiano, da parlamentare, ed anche da amante della storia del nostro straordinario Paese. Non mi soffermerò certo certo sulla storia che ha portato all'Unità d'Italia. Non lo farò perché lo si è già fatto abbondantemente ieri durante la discussione generale, e ne ha parlato anche stamani, in modo egregio, da par suo, il senatore Pardi, unendo letteratura e storia. Ma non posso non sottolineare un pizzico di amarezza per le tante polemiche che hanno portato poi a condividere questa festa nazionale dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Un pizzico di amarezza per coloro che non hanno compreso - e sono pochi - come il federalismo non sia alternativo all'unità, ma come, anzi, sia una componente essenziale per l'unità del Paese. Come ha ben detto il come si può pensare di far crescere il nostro Paese, se non cresce contemporaneamente il Mezzogiorno? Non si è compreso questo, e si è polemizzato anche su una cosa così scontata come la festa della nostra Unità, a distanza di 150 anni. Non guardiamo al passato, ma la memoria degli eventi che condussero alla nascita dello Stato nazionale unitario e la riflessione del lungo percorso compiuto successivamente possono risultare preziose per il momento difficile che attraversa il nostro Paese. È un momento estremamente complesso per il nostro Paese. L'unificazione italiana ha rappresentato un'impresa storica straordinaria per le condizioni in cui si svolse, per le che la accompagnarono e per i molti che sacrificarono la vita per questa unità. A partire da quel giorno, l'Italia afferma a voce alta la propria indipendenza e la propria libertà davanti al mondo intero. Sono d'accordo con il senatore Viespoli quando parla di un patto nazionale che preveda la crescita di tutto il Paese: non di una parte, ma di tutto il Paese, insieme ed unito. Mentre il senatore Viespoli ricordava una parte critica del discorso straordinario del Presidente della Repubblica, a me piace ricordare un momento bello di quelle parole, quando il Presidente della Repubblica ha detto: «Valgano dunque le celebrazioni del centocinquantenario a diffondere e approfondire tra gli italiani il senso della missione e dell'Unità nazionale». ci riusciremo ad una condizione: che operi nuovamente un forte cemento nazionale unitario, non eroso e dissolto da cieche partigianerie, da perdite diffuse del senso del limite e della responsabilità».

Signor Presidente, signori senatori, rappresentante del Governo, vorrei fare alcune brevi premesse e poi alcune considerazioni. Inizialmente, sul testo originale del provvedimento, il ministro Calderoli in Consiglio dei ministri aveva evidenziato come la copertura finanziaria fosse sbagliata; e aveva ragione a non votare un provvedimento con una copertura sbagliata. Fatto sta che in fase di valutazione del testo sono state apportate le modifiche necessarie a sistemare questa incongruenza. Ringrazio il relatore, senatore Pastore, per il lavoro certosino che ha svolto. Seconda Seconda premessa: siamo di fronte ad un decreto che nella sostanza conferma la legittimità di una festività goduta. Negare questa evidenza implicherebbe una serie di situazioni del tutto illogiche, comprese incresciose quanto evidenti ricadute sui lavoratori dipendenti. Quindi, per senso di responsabilità, viste le correzioni e le modifiche, la Lega Nord non si opporrà alla conversione del decreto. Detto questo, ritengo che la libertà di pensiero sia il sale della democrazia e a noi piace poter esprimere serenamente le nostre idee rispettando quelle degli altri, ma con umiltà chiediamo che anche gli altri rispettino le nostre. Lasciati alle spalle il 17 marzo e le quattro giornate delle celebrazioni dedicate al centocinquantenario, possiamo agevolmente constatare quanto abbiano trovato rispondenza nei fatti certe perplessità da noi avanzate. Non pensiamo soltanto al ponte vacanziero che c'è stato, riflesso condizionato della festa infrasettimanale, e alle sue ricadute economiche, ben poco consone al momento di crisi; ma ci riferiamo soprattutto all'altrettanto preannunciata strumentalizzazione dell'evento, previsione concretizzata da quanti, nell'anniversario dell'incoronazione del primo Re d'Italia, hanno agitato il Tricolore come una clava,

ricorrenza. Credo che a costoro sfugga un dettaglio: il Tricolore di oggi, secondo noi, anche formalmente, non è più quello della Real Casa, non è l'infausto drappo sventolato - lo ricordava il senatore Pardi - dalla soldataglia di Bava Beccaris, che rispondeva coi cannoni ai milanesi scesi in piazza a chiedere pane; non è l'insegna degli esattori reali che taglieggiavano con la tassa sul macinato i nostri contadini, condannandoli alla miseria e alla morte di pellagra; non è il sudario sui cadaveri dei ragazzi mandati a morire in sciagurate guerre coloniali; non è stendardo d'oppressione. No, il Tricolore d'oggi è la bandiera di uno Stato che ha cambiato il Titolo V della Costituzione attribuendo valenza federale alle Regioni, e che ha approvato il federalismo demaniale e il federalismo comunale già premono federalismo provinciale e regionale, nel contesto di un federalismo fiscale che è federalismo *tout court*: l'Italia del centocinquantenario diviene pienamente federalista. Conviene che certi improbabili garibaldini se ne facciano una ragione e comincino a guardare al Tricolore non più come al drappo savoiardo ma come alla bandiera di uno Stato federale.

persino a Garibaldi gli storici attribuiscono convinzioni federaliste, mentre un esplicito anelito federalista, anche spinto, direi confederale, appare negli scritti dei pensatori risorgimentali (la senatrice Adamo li ha ricordati nella discussione generale: questo dimostra che siamo anche attenti a quello che dite), come Cattaneo, Gioberti, Rosmini, Ferrari e Montanelli, per non parlare del "grande tessitore", quel Cavour che vagheggiava di tre Stati nella Penisola, uno al Nord, uno al Centro e l'altro al Sud. Ma su tutti prevalse la sete di potere di un sovrano e gli interessi di una oligarchia senza scrupoli, e fu la scelta centralista. È questo che anche noi avremmo dovuto festeggiare il 17 marzo? O forse, contestualmente all'incoronazione di Vittorio Emanuele II Re d'Italia, celebrare la nascita di un Parlamento che, su una popolazione di 26 milioni di abitanti, accordava il diritto di voto ad appena 400.000 cittadini, i più ricchi e i devoti dipendenti statali? Il presente ci mostra motivi più apprezzabili di festosità. Con le riforme avanzate e portate a buon esito con il contributo della Lega Nord, il Paese esce dal centralismo sabaudo e cresce; una Nazione adulta può anche fare i conti con il proprio passato senza nascondersi nel fumo della retorica. Nel caso di altri eventi storici, si è infine giunti ad ammettere il diritto alla memoria della parte soccombente. Perché il rispetto che si è accordato ai ragazzi di Salò viene negato a chi, nel periodo risorgimentale, ad esempio, stava dalla cosiddetta parte sbagliata? Il Regno Lombardo-Veneto, ad esempio, contava 60.000 uomini tra soldati ed ufficiali, lombardi e veneti, convinti di servire la loro patria e l'impero austriaco: compito che assolsero con onore, tanto che nel terribile teatro della battaglia di Solferino meritarono ben 112 medaglie al valore per atti di eroismo. Non minore ardimento dimostrarono i marinai veneziani a Lissa, quando al grido di «viva San Marco!» inflissero una clamorosa sconfitta alla neonata flotta italiana. Ed è con sincera commozione che penso alle decine di migliaia di militari del Regno delle due Sicilie, deportati in autentici *lager ante litteram*, da cui ben pochi uscirono vivi. Concludo, signor Presidente, sottolineando, se ce ne fosse bisogno, che non è per datato nostalgismo se ricordo gli esclusi dalla rimembranza ufficiale: il mio pensiero li comprende poiché sogno un Paese dove non si celebri un giogo centralista vecchio di 150 anni, bensì si celebri l'unione di intenti che scaturisce dalla libertà e dal rispetto di quello che ciascuno dei nostri popoli fu in passato, è adesso e sarà in futuro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, 12 anni fa, appena salito al Quirinale, il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in una condizione all'inizio di splendida solitudine, iniziò una tenace, martellante, convinta azione per valorizzare gli elementi fondanti della nostra Repubblica, del nostro Paese, della nostra Storia.

della bandiera, che veniva esposta quasi esclusivamente nel corso delle manifestazioni sportive e delle partite di calcio della Nazionale, e che tornò ad essere, giorno dopo giorno, sempre di più un modo in cui tornare a sentirci italiani. Continuò con la valorizzazione dell'Inno di Mameli, sino ad arrivare di nuovo a fare quello che molti cittadini di altri Paesi fanno: a cantare in tutte le occasioni pubbliche l'Inno del Paese. Carlo Azeglio Ciampi

i disagi, le speranze delle comunità locali, e cercando con la sua azione di Presidente della Repubblica, avvalendosi di tutte le sue prerogative, di valorizzare gli elementi della diversità, ma anche dell'unità del Paese. Chi come me, e come molti colleghi presenti in quest'Aula, ha svolto una funzione di amministratore locale, sa perfettamente che l'orgoglio dell'identità è un elemento essenziale per riprendere la strada della ripresa e della crescita di una comunità. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, da quattro anni, ha proseguito con il suo stile e la sua personalità esattamente la stessa identica azione: la valorizzazione dell'orgoglio della comunità del Paese e la ricostruzione puntigliosa della storia, in tutti i suoi chiari e in tutti i suoi scuri.

C'era un'aria di festa nelle strade della città. Ho visto la città piena di cittadini che avevano voglia di festeggiare questa giornata; la stessa identica cosa è avvenuta Firenze, pavesata da centinaia e centinaia di bandiere; la stessa cosa a Torino e nelle realtà del Sud del Paese. Una sensazione straordinariamente intensa di festa, che testimonia quanto lungimirante fosse stata l'idea del presidente Ciampi e poi del presidente Napolitano di andare in questa direzione. Voglio ricordare ai colleghi quanto è stato emozionante quando il presidente emerito Ciampi è entrato, sofferente, nell'Aula di Montecitorio accolto da un applauso da parte di tutto il Parlamento nei confronti di una personalità di eccezionale valore e di grande sensibilità.

e quando lo abbiamo intonato alla fine del discorso di Napolitano, quando la Banda Interforze aveva smesso di suonare e, spontaneamente, tutti insieme abbiamo intonato l'Inno di Mameli. Gruppo* *PD).* Penso che vada colto questo messaggio che il Paese ci dà: è un messaggio che supera i dubbi, le perplessità, i timori, se non addirittura la titubanza, di quelle forze politiche, anche della maggioranza, che sicuramente hanno sentimenti di forte orgoglio nazionale, ma che, sotto la pressione psicologica di non subire il distinguo della Lega, erano erano pronti a mettere da parte l'esigenza di manifestare intensamente questa giornata di festa; un messaggio che supera altresì la titubanza, le prudenze e i sottotoni che si sono registrati in questa occasione.

certamente ciò è possibile in un modo diverso e nuovo rispetto alla Costituzione originaria; è possibile anche grazie al fatto che la maggioranza degli italiani ha detto sì a quella riforma del Titolo V della Costituzione, che noi abbiamo voluto e che alcuni colleghi in quest'Aula non hanno votato!

Il Presidente del Consiglio rifugge tutte le occasioni in cui dovrebbe essere protagonista, nocchiero del Governo; in tutti i momenti difficili, egli scompare, e preferisce apparire con messaggi televisivi registrati, come si usa nelle peggiori dittature. troppo difficile parlare di fiducia in un momento in cui il Governo non si mostra all'altezza della situazione.

copertura economica: anche se le feste non hanno una copertura a livello di bilancio dello Stato, hanno un'incidenza particolarmente forte sull'economia. Si è tenuto conto di questa problematica e si è riusciti, attraverso il testo così ben spiegato dal senatore Pastore, a non creare ricadute negative. è stata anche l'intelligente obiezione del senatore Ichino, alla quale il collega Pastore ha dato una risposta riconosciuta congrua dallo stesso senatore che

Quando pensiamo a celebrazioni di questo tipo, abbiamo sempre il timore che prevalga l'aspetto retorico.

dell'essere pronti a donare la propria vita in ragione di un ideale. Io che sono di provenienza

Ma l'amore per la storia bisogna in qualche modo continuare a tenere vivo, come un prato che bisogna innaffiare spesso.

che fanno parte di un determinato contesto risorgimentale e ci fanno capire il sacrificio di Carlo Pisacane

Giovanni Ruffini, dovette emigrare in Inghilterra, dove scrisse il famoso «Il dottor Antonio», che sull'episodio risorgimentale incantò i lettori inglesi, tanto che il nostro Ponente ligure

interessano a tutti i livelli. Quando noi pensiamo a quello che il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio hanno portato avanti in queste celebrazioni, conto che hanno posto in essere punti importanti di riscoperta della cultura. Il «Nabucco» non è una delle grandi opere di Verdi; non è «Rigoletto», non è «Il Trovatore», non è «La Traviata» né «Otello»;

Non parliamo de «I Vespri siciliani», altra opera con una bellissima *ouverture*, benché tutto sommato non appaia tra le memorabili.

all'interessamento del nostro Presidente della Repubblica e del nostro Presidente del Consiglio rispetto

Visto il tema in discussione, credo che ciò abbia un particolare significato.

Il modo migliore per festeggiare l'unanimità sul voto precedente è ora quello di continuare a lavorare con serietà e in modo dignitoso. È questo il modo vero,

il dissesto idrogeologico, la tutela penale dell'ambiente, la gestione corretta dei ciclo dei rifiuti e le fonti energetiche rinnovabili. Argomenti che riteniamo fondamentali per una strategia di indirizzo politico su temi in cui vedevamo e vediamo ancora oggi una preoccupante carenza di iniziativa del Governo.

Presidente. È evidente a tutti come un Paese moderno e industrialmente avanzato quale l'Italia vuole essere debba dotarsi di un quadro energetico di indirizzo e di programmazione che abbia come obiettivi, a breve e a lungo termine, la diversificazione delle fonti di energia e delle aree di approvvigionamento, la promozione delle fonti rinnovabili, il risparmio e 1'efficienza energetica, la valutazione del fabbisogno nazionale e, conseguentemente, la programmazione delle tipologie di impianti necessari. È chiaro che nel predisporre un programma energetico non si può non tener conto anche del quadro di riferimento internazionale. L'andamento dei prezzi, la disponibilità delle fonti, le criticità geopolitiche sono elementi che nessun Governo può trascurare. Ma un ulteriore ed imprescindibile requisito è il riferimento alla normativa comunitaria di settore, che ha tra i suoi principali obiettivi la sostenibilità ambientale, il potenziamento della ricerca e dell'innovazione nella produzione energetica. Dobbiamo allora chiederci quale sia stata finora la strategia seguita dal Governo italiano. Se analizziamo i provvedimenti legislativi riguardanti le fonti rinnovabili, possiamo certamente concludere che una strategia non c'è. Questa maggioranza prima ha deciso di stravolgere il sistema di incentivi vigente, che aveva innegabilmente bisogno di aggiustamenti e correzioni; poi, dopo essere intervenuta con l'accetta, si è assunta l'impegno di ricucire le ferite causate ripristinando sostanzialmente quanto già previsto. Nel frattempo, però, il Governo ha portato avanti una accelerazione del programma nucleare, in palese controtendenza sia rispetto alla situazione internazionale, che vedeva un arretramento del nucleare già prima dell'incidente alla centrale giapponese, sia rispetto alla necessità di investire nelle rinnovabili. In realtà, quindi, l'unica strategia di questo Governo è stata quella di soffocare nella culla le rinnovabili e puntare tutto sul nucleare. Ma non possiamo più permetterci, in questo campo, errori così grossolani: è arrivato il momento di porvi rimedio. La moratoria sul nucleare che il Governo ha stabilito, sull'onda dei sondaggi sfavorevoli, non costituisce un ravvedimento significativo. Ma ci penseranno i cittadini italiani, siamo sicuri, con il *referendum*, ad eliminare dall'orizzonte dell'Italia i rischi generati da una fonte energetica così pericolosa, impattante, costosa, ambientalmente e territorialmente non sostenibile. Invece, a rimettere ordine nel settore delle rinnovabili potremo provvedere da subito in Parlamento, oggi stesso, indirizzando il Governo su quella che potremmo chiamare la retta via. A dire la verità, che si stesse prefigurando un pasticcio nel recepimento della direttiva sugli incentivi alle rinnovabili il nostro Gruppo Italia dei Valori del Senato lo aveva compreso da tempo, non votando a favore di quel parere parlamentare debole e contraddittorio che poi persino il Governo ha disatteso, aggravando la confusione del settore. quindi bene che ora al Senato, dopo la Camera, si ritrovi un comune sentire sulle correzioni da apportare al decreto governativo. La nostra visione sul ruolo delle fonti rinnovabili è chiara: si inserisce in una concezione dell'autonomia energetica nazionale che non offre spazio ad impianti nucleari dal costo esorbitante e dai rischi elevatissimi, che potrebbero coprire, se mai fossero attivate almeno due centrali entro il 2020, neppure il 5 per cento del fabbisogno interno. Mentre ci attardiamo su un nucleare che accrescerà la dipendenza energetica e tecnologica dall'estero, stiamo trascurando il fatto che le fonti alternative pulite, accusate a sproposito di non competitività, vanno avanti a ben altro ritmo.

in particolare, che ha una esposizione al sole infinitamente inferiore al nostro Paese, per motivi geografici e climatici che tutti conosciamo, surclassa l'Italia in campo solare. E la Germania non è notoriamente un Paese in cui si dilapidano soldi in meccanismi inefficienti: non a caso aveva deciso, già prima dell'incidente di Fukushima, di uscire dal nucleare puntando a soddisfare nel 2050 almeno l'80 per cento della richiesta elettrica con le rinnovabili. In risposta ai programmi di incremento delle fonti rinnovabili, attivi in diversi Paesi europei, il 2009 ha confermato la tendenza del decennio: le fonti rinnovabili hanno ampiamente superato le altre tecnologie di produzione dell'energia in termini di nuova capacità produttiva (ben il 62 La tecnologia eolica, nel 2008, è stata la fonte energetica con maggiore capacità produttiva annua, installata nell'Unione europea; primato che si è ripetuto nel 2009. Al pari di quella eolica, anche l'energia solare ha fatto riscontrare una enorme crescita nella capacità generativa installata. Il progetto solare termodinamico Desertec dovrebbe coprire a regime

pregiudizialmente contraria alle fonti fossili, prevede che nel 2030 la quota delle rinnovabili nell'offerta di energia avrà superato quella del nucleare. L'elettricità producibile dagli impianti solari ed eolici installati nel mondo tra il 2005 e il 2010 è tre volte maggiore rispetto a quella dei reattori nucleari entrati in servizio negli stessi anni. La metà della potenza elettrica installata in Europa è rinnovabile. La potenza fotovoltaica globale installata nel 2010 è, ad esempio, aumentata del 120 per cento rispetto all'anno precedente. dunque dubbio alcuno sulla necessità di non rimanere tagliati fuori da questo mercato. Ed il primo passo da compiere è quello di tornare ad offrire agli operatori, ai cittadini, alle istituzioni, quelle certezze che il recente decreto legislativo sulle rinnovabili ha malamente eliminato. Si può discutere su quanto gli incentivi pesino sulle bollette dei cittadini che li finanziano, ma la questione dovrebbe essere considerata alla luce degli obiettivi di diffusione delle rinnovabili e di sviluppo di una filiera industriale tecnologicamente avanzata all'interno del Paese. L'energia verde costituisce un comparto che impiega direttamente tra i 25.000 e i 30.000 lavoratori, tra cui un numero elevato di ingegneri, professionisti e tecnici specializzati, ovvero occupazione qualificata in buona parte localizzata al Sud, che raggiunge, con il lavoro indiretto dell'indotto, le 100.000 unità e che presenta tassi di crescita dell'occupazione superiori a tutti gli altri settori dell'economia italiana, elemento non da poco in una fase di congiuntura come quella attuale. Riflettere sui meccanismi più efficaci per il sostengo all'industria delle rinnovabili, lo ribadisco, è del tutto legittimo per un Paese che ha assunto nei confronti dell'Unione europea e delle future generazioni l'impegno di produrre energia in modo indipendente dal petrolio e non inquinante. Andrebbe però fatto con razionalità, nei modi e nei tempi opportuni. Non si possono fare provvedimenti retroattivi, non si può dire: «Abbiamo scherzato, ora cambiamo tutto». Soprattutto, non si può legiferare sotto la pressione di interessi potenti o sotto la pressione di campagne di informazione fasulle. Per questo nella nostra mozione chiediamo di attuare una strategia coerente, stabile ed organica di potenziamento delle fonti rinnovabili pulite. Chiediamo di rivedere i meccanismi di incentivazione nel senso di favorire l'innovazione tecnologica, la trasparenza delle procedure e la garanzia degli investimenti effettuati. Chiediamo la riduzione del carico sulla bolletta elettrica, oggi impropriamente destinato a beneficio delle cosiddette fonti assimilate CIP6. Chiediamo al Governo di emanare i provvedimenti correttivi in materia di definizione del quantitativo incentivabile. Ovviamente è indispensabile un parallelo abbandono del programma nucleare. Ma il secondo passo da compiere è quello di eliminare alcune storture che in passato si sono verificate nella gestione concreta del mercato dei certificati verdi. Non si vede perché Germania e Austria, che puntano sulle rinnovabili, non conoscano quelle patologie che noi riscontriamo in Italia. Ci sono state inchieste della magistratura che hanno aperto squarci preoccupanti

in modo da produrre energia in una misura più integrata al paesaggio ed alla specifica storia e tradizione locale, procedendo d'intesa con le soprintendenze regionali e di settore e sempre secondo logiche di utilità pubblica. Per questo è cruciale il coordinamento e l'integrazione tra il contenuto dei piani nazionali e regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici, con il fine di perseguire gli obiettivi di produzione da fonte rinnovabile definiti dall'Europa.

mantenere, anche nei toni, un atteggiamento costruttivo, che mira a risolvere un problema. parlare, seppur rapidamente, della storia che ci ha portato a questo punto e a questa giornata che il Senato dedica alle energie rinnovabili. Tale storia è

in particolare, avevamo apprezzato che in quel decreto sulle rinnovabili si affrontasse finalmente la questione relativa al

tranne per alcuni punti fondamentali del decreto che correvano il rischio di inficiarne la positiva ispirazione. Nel percorso parlamentare, sia qui al Senato sia alla Camera, Camera, in condivisione con la maggioranza abbiamo provato a correggere quegli aspetti negativi, tant'è che il parere poi reso dalla Commissione competente è stato votato all'unanimità con una serie di condizioni che non sto qui a ripetere, anche perché le più rilevanti sono riportate solo un esempio. Un punto essenziale che ponevamo come condizione per l'approvazione del decreto riguardava il sistema che, a regime, dovrebbe regolare le incentivazioni, e che il Governo prevede essere di aste al ribasso.

ricorso fosse elevato, rispetto ai soli cinque megawatt previsti dal Governo. Nonostante questo percorso positivo, lo ribadisco, che ha portato all'approvazione all'unanimità dei pareri, sia alla Camera che al Senato, il Governo, nell'emanazione definitiva del decreto, non solo non ha ritenuto di tener conto delle condizioni più rilevanti che gli avevamo posto come Parlamento, ma ha fatto peggio, cioè ha introdotto in maniera del tutto improvvida e imprevista, perché nessuno glielo aveva chiesto prima, un intervento sul fotovoltaico, peraltro non previsto nella versione originale del decreto, che ha portato ha portato a un blocco totale degli investimenti su questa tecnologia dal 3 marzo a oggi. Se a ciò si abbina il fatto che le aste, come dicevo prima, si svolgono con un sistema piuttosto complicato, che coinvolge anche l'eolico,

importante che nel decreto attuativo del decreto legislativo attualmente in discussione, su cui si stanno svolgendo, per quanto ne sappiamo, anche dei tavoli tecnici,

un elemento criminale, che invece noi vogliamo evitare, perché siamo tutti contro le speculazioni. Quindi, nessun tetto. Si pensi, piuttosto, a un sistema tedesco per cui la soglia

sempre tenendo conto però degli equilibri tra il miglioramento tecnologico che permette la diminuzione delle tariffe incentivanti e tariffe che siano però sostenibili per permettere gli investimenti necessari. Dal momento, poi, che sappiamo

pensare ad un tetto economico sulla tariffa A3 che riguardi tutte le energie rinnovabili e, in base a quello, modulare gli incentivi in modo che ogni settore abbia la sua convenienza.

per il fatto che non siamo riusciti a realizzare il cavo di collegamento fra la Sicilia e la Calabria. Potrei continuare con tante altre spese inutili e improduttive che pesano oggi sul costo dell'energia e che, contrariamente alle energie rinnovabili, sono

certezza nel futuro a un settore così importante per il nostro Paese.

alle recenti dinamiche geopolitiche nell'area del Mediterraneo che, purtroppo, non ci fanno stare molto tranquilli. Il nostro Paese è notoriamente da sempre un importatore di energia (gas, petrolio, carbone)

Tutto questo anche in conseguenza del fatto che l'Italia ha dismesso, purtroppo, da oltre vent'anni le proprie centrali nucleari,

dal punto di vista economico nel nostro Paese, visto che oggi - come dicevo prima - siamo quasi totalmente dipendenti dall'estero in quanto ad approvvigionamento di risorse energetiche. Negli ultimi anni

economico generato dalle energie rinnovabili nel nostro Paese: un indotto che negli anni è arrivato a dare occupazione a più di 150.000

È per questo che con giustificata preoccupazione abbiamo appreso dell'ultimo decreto del Ministro, un decreto che non disegna un futuro molto roseo alle energie rinnovabili nel nostro Paese. Siamo convinti - e concordiamo con il Ministro - che serva fare chiarezza sul fatto che le energie rinnovabili non gravino troppo sulla nostra bolletta elettrica. Siamo ancora più convinti del fatto che investire sulle rinnovabili è investire sul futuro dei nostri figli. Con questa mozione il Gruppo della Lega Nord chiede siano ascoltate le richieste dei tanti operatori e investitori del settore, che incontrano sicuramente anche il parere positivo di tutti o della stragrande maggioranza dei cittadini del nostro Paese, Paese, all'unico scopo di dare un futuro a questo settore e alle tante persone che ci lavorano. Chiediamo che quanto prima sia emanato - e mi pare che sia in corso di definizione - un nuovo decreto che vada appunto in questa direzione, ponendo fine all'attuale situazione di incertezza che provoca solo disagio ai lavoratori, agli investitori e a tutti quei cittadini (e sono tantissimi) che credono che le rinnovabili siano o possano essere il punto di partenza per un ambiente e un futuro migliore per il nostro Paese. Chiediamo vengano mantenuti i benefici della norma introdotta su proposta del nostro Gruppo, la Lega Nord, nella legge n. 99 del 2009, norma molto apprezzata ed utilizzata dai sindaci, con cui si dà la possibilità ai Comuni di autoprodursi l'energia elettrica fino a una potenza di 200 chilowatt, con notevole beneficio ambientale ma anche per le casse dei Comuni. Chiediamo, in attesa che venga definita la questione del nucleare, che non si abbandonino ma che si incentivino le energie rinnovabili, le uniche forme di energia che usano la forza della natura contribuendo sicuramente e fortemente a salvaguardare l'ambiente, e credo sia giusto giusto ricordare gli obiettivi che il nostro Paese si è prefissato con il pacchetto clima-energia, il famoso obiettivo 20-20-20, finalizzato a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra.

Governo per addivenire ad una soluzione unitaria e condivisa non soltanto tra i Ministeri, ma anche tra gli operatori del settore, tra le associazioni, stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo dove i Ministeri interessati, le associazioni e gli imprenditori di categoria siedono tutti insieme affinché entro il 30 aprile si definisca una certezza sul quadro normativo legato proprio agli incentivi nel settore delle rinnovabili. Questo è un fatto importante, che deve darci una speranza in più, ci deve incoraggiare a sostenere questo lavoro, perché riuscire a dialogare tutti insieme è un fatto certamente di grande serietà e certezza di arrivo al punto che tutti quanti desideriamo. Voglio anche ricordare che in questo senso la Commissione industria del Senato, con tutte le sue componenti politiche, ha lavorato dalla fine dell'anno scorso sino a qualche giorno fa definendo un parere condiviso non soltanto dalla maggioranza ma anche voglio sottolineare - dal Partito Democratico; parere che è nato dopo due mesi e mezzo circa di lavoro e dopo ben 33 audizioni che sono state svolte dalla Commissione avendo sentito direttamente dai destinatari delle delle misure tutte le problematiche connesse. La mozione che oggi viene qui presentata raccoglie un po' tutto questo lavoro e, in sintonia con il Governo, credo che le proposte che - mi auguro - dal Parlamento possano trovare accoglimento nei futuri decreti attuativi che il Governo dovrà adottare. Voglio anche far presente che l'Agenzia internazionale per l'energia

di una riduzione delle fonti primarie di energia. In questo quadro emerge una chiarezza nella nella certezza di intervento per fronteggiare un aumento non soltanto dei consumi, così come vi dicevo, ma anche di quanto è legato ai consumi, cioè le emissioni di CO2. Per questo motivo è necessaria una politica che incentivi e dia certezza normativa nel settore delle rinnovabili, considerando che la dipendenza dalle fonti fossili

entro il 2020 del 17 per cento di energia prodotta nel settore delle rinnovabili e del 10 per cento di energia verde nei trasporti.

è andato avanti. Anche la strategia energetica nazionale del nostro Paese ci aiuta in tale percorso e ci indica delle priorità

la promozione delle fonti rinnovabili; soprattutto - lo voglio ricordare - l'efficienza energetica. Senza una grande sensibilità e un forte impegno da parte del Governo, ma soprattutto dei clienti finali, a comprendere che non dobbiamo soltanto chiedere di poter usare tutto ciò che vogliamo, ma che occorre sviluppare una capacità di risparmio dei singoli destinatari di questi provvedimenti, ossia individui e famiglie, i nostri sforzi verranno resi assolutamente vani. Sul tema dell'efficienza energetica e del risparmio energetico forse dovremo fare ancora qualche sforzo in più.

La scelta, a questo punto, non può essere legata esclusivamente ad un problema nazionale, ma ad un problema europeo sul tema nucleare.

alcuni punti che sono stati a lungo dibattuti in Commissione e ripresi nella mozione: l'accelerazione dei tempi per la definizione puntuale dell'incentivazione all'evoluzione del fotovoltaico e dei biocarburanti, punto inserito nel parere e ripreso nella mozione, chiarendo in modo assolutamente trasparente l'impatto dei costi degli incentivi sulla bolletta elettrica; il raggiungimento della *grid parity* e delle misure volte a contenere i tempi di allaccio alla rete (anche su questo si dà certezza all'investimento); la previsione di un *floor* minimo, a seconda del tipo degli impianti, nel meccanismo nel meccanismo dell'asta al ribasso. Questi secondo noi sono punti che devono essere tenuti in considerazione e mi auguro che il Parlamento nella sua composizione possa accoglierli, così come anche noi condividiamo

Governo: il decreto del 3 marzo scorso, relativo agli incentivi sul fotovoltaico, e la moratoria sull'individuazione dei siti per le centrali nucleari.

ma dobbiamo anche dire che non possiamo ripetere gli errori del passato: nel 1987, a seguito dell'incidente di Chernobyl dell'anno precedente, l'Italia rinunciò al nucleare; tutti gli altri Paesi, che sento citati in quest'Aula come virtuosi, hanno viceversa continuato a sviluppare questa attività, diventando anche esportatori. È il caso della Francia, che con i suoi 58 impianti permette all'Italia di avere l'energia sufficiente al proprio fabbisogno;

dove viene peraltro sviluppata una ricerca straordinaria per il futuro, che è quella della fusione nucleare con l'impianto Kadarash, sito in una delle zone più belle della Provenza e della Francia.

il terremoto in Giappone e la crisi dell'impianto giapponese di Fukushima. L'emotività delle popolazioni anche europee,

tentare di decidere non «di pancia», ma razionalmente, pensando agli interessi della nostra Nazione e dei nostri concittadini. Apro una breve parentesi su quanto è avvenuto proprio a Fukushima. Rispetto ad una emotività enorme che ha attraversato il globo, ricordo a quest'Assemblea che non vi è stata una sola vittima (è un conto cinico e bruto

Credo dunque che, contestualizzando tale emotività, possiamo accettare il provvedimento del Governo, ma dobbiamo ricordarci che il futuro non può non mettere in conto questo tipo di attività, perché è la sola che

Recentemente è stata pubblicata dalla rivista specializzata «Edilizia e Territorio» una tabella che confronta la situazione italiana con quella di altri Paesi europei come Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Il confronto è impietoso e testimonia come il valore degli incentivi in Italia sia il più elevato. Infatti, oltre al valore degli stessi, vi è la possibilità di sommare ad essi il *premium,* ovvero la vendita di produzione elettrica. È evidente che tale sistema (come accertato dal Ministero delle attività produttive e dallo stesso ministro Romani), di fronte ad una crescita esponenziale degli impianti solari e fotovoltaici,

decidere un intervento imperativo per regolamentare e rimodulare il sistema. Non dobbiamo dimenticare che l'obiettivo previsto nella direttiva dell'Unione europea europea conosciuto con la sigla 20-20-20, all'interno del quale l'Italia aveva previsto di realizzare 8.000 megawatt entro il 2020, secondo secondo i numeri oggi conosciuti sarebbe raggiunto entro il 2012. Pertanto, mentre riteniamo assolutamente da condividere la proposta del Governo, con il decreto del marzo scorso relativo alle correzioni delle distorsioni risultanti dalla nostra normativa in aggiunta a quelle testé specificate, bisognerebbe anche ricordare la necessità di bloccare la speculazione su questo tipo di attività, che si era fortemente sviluppata in virtù degli incentivi, ma anche di una estrema semplificazione delle procedure autorizzative su base regionale e di una estrema diversificazione. Per questo noi riteniamo, con la mozione in esame, di indicare al Governo una soluzione affinché il termine imperativo del 31 marzo prossimo, previsto dal citato decreto - data entro la quale potranno accedere agli incentivi correnti soltanto gli impianti allacciati - debba essere corretto, in virtù del fatto che gli interventi autorizzati hanno un *iter* di realizzazione significativamente lungo, che l'allaccio non dipende dalle imprese ma dall'ENEL e che il controllo del GSE è molto lento. Per quanto ci risulta, su 3.954 megawatt dichiarati nel 2010, il GSE ne aveva controllati, al 28 febbraio scorso, soltanto 338. Chiediamo pertanto al Governo di dare stabilità al quadro regolatorio, salvando intanto gli operatori che hanno già in mano l'autorizzazione.

credo che per ogni Governo, e soprattutto in questo particolare momento della nostra storia, la questione dell'energia, e quindi il problema dell'approvvigionamento energetico, sia davvero molto delicata e importante. Ritengo anche che la questione energia sia un asse strategico che ogni Governo di buon senso dovrebbe inserire a livello prioritario nel suo programma, perché da essa dipende poi la possibilità dello sviluppo del Paese e della qualità della vita dello stesso.

Grazie e sugli utenti. Tutto ciò che è accaduto, infatti, sulla questione dell'energia - che va vista in maniera ampia e soprattutto articolata così come ci ha indicato l'Unione europea sta ad indicare che ad oggi non ci sono, né idee chiare, né certezze, così come avvenuto per quanto riguarda la

situazione contingente e quindi dall'emergenza che si sta vivendo, con tutti i riflessi emotivi che comporta, se vogliamo portare avanti una decisione consapevole, e soprattutto mirata ad una qualità della vita e allo sviluppo del nostro Paese, a meno che non vogliamo tornare a tempi molto lontani, nei quali non c'era stato il processo di industrializzazione, si viveva in maniera diversa e vi era un minore bisogno di energia. è vincolante per qualsiasi mossa che si faccia sullo sviluppo economico; l'energia è vincolante anche per la qualità della nostra vita, per la ricerca scientifica e tecnologica; è un qualcosa di cui non possiamo fare a meno. È chiaro però, così come ci ha detto l'Unione europea, che dobbiamo prevedere dei limiti e limitarci rispetto alla capacità, dovuta al consumo di energia, di continuare a immettere

Dobbiamo soprattutto eliminare quel quantitativo di sostanze tossiche che immettiamo nell'atmosfera attraverso una politica che riequilibri le fonti energetiche, puntando anche sulle energie rinnovabili.

i nostri terreni agricoli e ha consumato il territorio in maniera inopinata e soprattutto non accettabile dal punto di vista della questione agricoltura, della produzione dei nostri prodotti più pregiati, quelli DOC per esempio. Le nostre colline, oltre a costituire un bene paesaggistico che va tutelato - come va difeso tutto il nostro patrimonio culturale e paesaggistico - sono anche da tutelare rispetto al problema della capacità di produzione agricola, che viene in qualche modo limitata e compromessa. C'è una distesa di pannelli al suolo che non è stata caratterizzata da una progettazione e una pianificazione attenta da parte delle Regioni e degli enti locali, tant'è, che di fronte a questo arrembaggio, e alla denuncia, anche da parte delle confederazioni agricole,

le società straniere. Negli altri Stati europei si è preceduto a limitare e a organizzare la questione delle rinnovabili e ad inserirla all'interno di dispositivi corretti, applicabili e soprattutto intelligibili da tutti;

La stessa *Authority* per l'energia sostiene che gli incentivi concessi al fotovoltaico sono tra i più profittevoli del mondo: il costo medio dell'energia si aggira tra i 60 e i 70 euro al megawattora

Rispetto alla direttiva comunitaria, l'Esecutivo oggi deve intervenire sul sistema normativo relativo agli incentivi per la produzione di energia, cercando soprattutto di frenare la speculazione nazionale e internazionale e cercando di non varare provvedimenti retroattivi che vadano anche a inficiare interessi legittimi che si sono instaurati:

che riguardano tali questioni in modo particolare, bisogna cercare di evitare un ulteriore rinvio per la regolazione della disciplina delle incentivazioni. che il decreto che il Governo si appresta ad adottare riesca a determinare in maniera chiara, leggibile e soprattutto onesta e trasparente, una legislazione che limiti, e addirittura elimini, l'incertezza normativa per tutti gli operatori che, sulla base delle disposizioni tuttora vigenti, hanno realizzato

perché la nuova disciplina non può prescindere da questo momento concertativo. Chiediamo che si promuovano anche un'attività di ricerca, che ci sembra indispensabile rispetto alle fonti rinnovabili, rinnovabili; a promuovere misure atte a disincentivare i comportamenti speculativi degli operatori, in particolare quelli orientati a realizzare investimenti esclusivamente orientati a logiche finanziarie;

Soprattutto chiediamo che vi sia una linea chiara del Governo rispetto alla questione energetica come asse fondamentale per la politica di sviluppo del nostro Paese.

la mozione di riferimento intende contribuire ad un ripensamento del Governo circa le sue più recenti decisioni in materia di fonti energetiche rinnovabili. Le premesse e gli impegni conseguenti sono in linea con altre e spesso più dettagliate considerazioni contenute nelle altre mozioni oggi in discussione e non richiedono un particolare, ulteriore approfondimento. I proponenti non intendono sostenere interessi di specifici gruppi di pressione, quanto piuttosto tentare un approccio ampio al tema dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, alla luce del deludente esito del confronto fra Governo e Commissioni parlamentari competenti in vista della adozione del decreto legislativo dello scorso 3 marzo 2011. Molte delle condizioni e delle osservazioni proposte allo schema di decreto legislativo non sono state assolutamente considerate: esempio preclaro di scarsa considerazione del Parlamento e, aggiungerei, della maggioranza, che in esso pur sostiene il Governo. Peraltro, le scelte sulle restrizioni alle incentivazioni, già presenti nelle normative di bilancio, così come, in settore connesso, il poco elegante cerchiobottismo sull'energia nucleare, palesato dalle recentissime decisioni del Consiglio dei ministri, sono lampi che rischiarano un panorama di incertezze, eretto a sistema nel comparto energetico. Cosa vuole il Governo, dove vuole portare l'Italia? È facile dire: tagliamo su tutto, risparmiamo su tutto, rispettiamo le direttive europee. Ma per quale prospettiva? Il nucleare è decisamente di là da venire là da venire sarebbe positivo sentire dal Governo una parola di chiarimento sulle opzioni francesi, sul loro costo, sugli impegni già assunti. Quanto stona l'irrigidimento verso la Francia sulla vicenda libica rispetto, per esempio, alla vicenda Alitalia, o a quella Parmalat o, appunto, a quella nucleare. Sull'eolico si proiettano le ombre della criminalità e della speculazione, senza che si prospetti un indirizzo normativamente accettabile sotto il profilo urbanistico-ambientale e sotto quello procedurale, con adeguato riferimento a Regioni ed enti locali per le rispettive competenze. Sul fotovoltaico si potrebbero dire le stesse cose, con l'aggravante che la confusione tra privati imprenditori e speculatori sta creando una grande incertezza di prospettive per i singoli (nuclei familiari, edifici residenziali) che non intravedono più la convenienza della opzione; mentre si dismettono - per uso improprio dobbiamo pur dire - parti significative di territorio, con l'aggiunta delle note problematiche circa i finanziamenti bloccati, le banche sospese e un mercato florido (e la connessa occupazione) sull'orlo della crisi. Considero scandalosa la omissione circa l'energia idroelettrica, primaria fonte rinnovabile, caratterizzante soprattutto l'area alpina, che chiede solo l'attenzione dovuta ad una necessaria - diremmo - e continuativa manutenzione degli impianti esistenti e in produzione, l'età media dei quali giustifica simili interventi e - per la peculiarità del fattore energetico acqua - giustifica ampiamente anche il conseguente incentivo. Anche in questo caso il rinvio alle audizioni (si leggano i verbali) e alle osservazioni (si leggano i pareri) delle Commissioni può bastare. Una compiuta attenzione del Governo al tema complessivo, traducibile in un deciso impegno di promozione - non formale - sia di una diversificazione ampia delle fonti rinnovabili (come avviene in altri Paesi europei) sia di una nuova cultura da indurre nella popolazione, certamente significa utilizzo di risorse pubbliche, la distorsione nella gestione delle quali non è motivo sufficiente per fermare la progressione del sistema. Anzi, lo stimolo ad una forte evoluzione italiana dell'intero comparto

al raggiungimento di obbiettivi di contenimento e di sviluppo, che - prima di essere aride sequenze in documenti internazionali - segnalano la capacità di innovazione e di effettiva evoluzione del nostro Paese. In queste prospettive vanno considerati, nel dettaglio, gli impegni indicati nella mozione.

mi auguro veramente che gli atti di indirizzo che oggi approveremo consentiranno di modificare e di rimediare al grave errore che il Governo ha compiuto in materia di energie rinnovabili. Quello che emerge più in generale è una grave inaffidabilità del Governo in materia energetica. Parlate di modifica dell'articolo 41 della Costituzione - fumisterie ideologiche - e in concreto alterate e turbate un intero settore economico, le decisioni di investimento, di imprese e famiglie: altro che articolo 41 come inciampo allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Voi siete il maggiore inciampo, con questi gravissimi errori.

inoltre bisogno di molta capacità della politica di offrire indirizzi chiari, permanenti e condivisi. Possiamo dire che questo Governo abbia costruito un quadro che vada in questa direzione rispetto ai due grandi pilastri alla base di una politica energetica, e cioè la diversificazione delle fonti e la riduzione dei consumi? Ricordo che abbiamo un PIL molto energivoro. Ogni punto di aumento del PIL significa un aumento dello 0,9 per cento dei consumi di energia elettrica. Bisogna agire su questo settore. Noi l'avevamo fatto con convinzione:

incentivi molto robusti per l'isolamento termico degli edifici. A tecnologia esistente, si calcola che si potrebbe ridurre del 30 per cento il consumo dell'energia. Avete completamente abbandonato queste politiche, o le avete indebolite. Per quanto riguarda la diversificazione delle fonti vi siete avviati su questo *spot* del nucleare. Non sono ideologicamente contrario al nucleare,

Informo i signori della maggioranza che ieri il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una mozione che dice no ad ogni insediamento di centrali nucleari. Come non capire che il nucleare è molto costoso dal punto di vista degli investimenti e che non è affatto vero che sia in espansione nel mondo? L'Agenzia internazionale dell'energia che negli ultimi dieci anni la componente nucleare nella produzione di energia elettrica è passata dal 17,2 al 14 per cento. Avete ignorato ogni avvertimento, e oggi, qual è la vostra affidabilità? Ricordo che avevate detto che entro l'autunno del 2009 (due anni fa) vi sarebbe stata l'individuazione dei quattro siti per le centrali di cui all'accordo con la Francia vi sarebbero stati i primi kilowattora prodotti dall'energia nucleare. È evidente che eravamo nel regno della fantasia. avete paura dell'opinione pubblica e proponete una moratoria, che è esattamente il contrario di ciò di cui ha bisogno il Paese, cioè chiarezza e certezza. Per affidarvi all'impossibile (il nucleare) non fate il possibile. Penso ad esempio a ciò che si potrebbe fare valorizzando la fonte idroelettrica, di cui parlava il senatore Molinari, quello che si può fare per mettere in sicurezza l'approvvigionamento del gas attraverso un piano serio di rigassificatori.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il tema dell'energia da fonti rinnovabili è da sempre strettamente legato agli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale ed europeo. Il Governo Berlusconi, fin dall'inizio della legislatura, ha dedicato particolare attenzione alla *green* *economy*, nella consapevolezza della necessità di ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera e di aumentare sensibilmente la propria quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Tutto questo ha consentito all'Italia di raggiungere importanti traguardi nel settore dell'eolico, del fotovoltaico e del geotermico. Questo importante sviluppo dell'energia verde ha sicuramente prodotto, negli ultimi anni, investimenti rilevanti che hanno generato nuova occupazione e, soprattutto, la nascita di piccole e medie imprese specializzate, ad esempio, nell'installazione di piccoli impianti per le famiglie. Le stesse famiglie italiane hanno contribuito a far crescere questo settore decidendo di avviare nelle proprie case interventi di riqualificazione degli edifici volti al risparmio energetico e all'installazione di pannelli fotovoltaici. Ora però dobbiamo riconoscere che questo importante settore è riuscito a svilupparsi, non solo grazie all'ingegno italiano e a tutti i cittadini che hanno veramente creduto di dover dare il loro contributo all'ambiente, ma anche grazie ad un sistema di incentivi che è stato sicuramente tra i più generosi d'Europa. Questi incentivi però, come tutti noi sappiamo, hanno gravato negli anni sulle bollette delle famiglie italiane e delle imprese, imprese che, oggi più che mai, debbono confrontarsi con una realtà globale sempre più competitiva. Il Governo, pertanto, ha avuto il coraggio di porre per la prima volta l'attenzione sul costo in bolletta di questi incentivi nel fare tutto questo, ha tenuto chiaramente presente il fatto che lo sviluppo tecnologico nel settore delle rinnovabili ha consentito, nel giro di pochi anni, di abbattere i costi per la realizzazione degli impianti. Tuttavia, nel perseguire questo obiettivo, senz'altro lodevole, non si può non tenere in considerazione la necessità di assicurare ad un comparto così strategico per l'intera economia nazionale dei meccanismi di gradualità.

riguardo, ha avuto la capacità di ascoltare le istanze degli operatori del settore e delle associazioni di categoria, trovando un giusto equilibrio tra la necessità, da un lato, di ridurre gli oneri in bolletta e, dall'altro, di salvaguardare gli investimenti programmati, sui quali, magari, erano stati concessi dalle banche i necessari finanziamenti alle famiglie e alle imprese. È anche per questo che oggi siamo qui in Senato a discutere di queste mozioni, che consentiranno al Parlamento di tracciare una rotta che, sono sicuro, il Governo seguirà. I primi segnali positivi tangibili si sono già avuti nei giorni scorsi, quando i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e dell'agricoltura hanno avviato un tavolo di confronto con tutte le realtà interessate e con gli istituti bancari che hanno erogato i necessari finanziamenti negli scorsi mesi. Tutto ciò, onorevoli colleghi, è sicuramente indicativo di come il Governo abbia ben compreso l'importanza di un confronto tra tutti gli attori, che, sono sicuro, nelle prossime settimane sarà proficuo e consentirà all'Italia di salvaguardare un comparto strategico e di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione Europea con l'adozione del cosiddetto pacchetto clima-energia. Il confronto di oggi tra Governo e Parlamento e le mozioni che ci accingiamo ad approvare daranno quindi

pacchetto clima-energia. Il confronto di oggi tra Governo e Parlamento e le mozioni che ci accingiamo ad approvare daranno quindi nuova fiducia agli investitori, alle imprese e ai cittadini italiani che da sempre hanno creduto nelle energie rinnovabili. *(Applausi dal

in un clima di grande, diffuso e crescente disorientamento nel Paese. Nelle ultime settimane, infatti, per ragioni così lontane, ma rese contestuali dagli eventi, abbiamo avuto: la crisi libica, che ha messo in discussione uno dei nostri principali canali di approvvigionamento di gas e petrolio; la tragedia giapponese, che ha prodotto nel mondo intero una profonda riflessione sulla scelta nucleare, costringendo il Governo italiano alla moratoria dell'annunciato ritorno al nucleare e la questione delle energie rinnovabili, di cui ci occupiamo oggi, messa in crisi dall'approvazione del decreto legislativo che sostanzialmente azzera gli incentivi, in particolare, per il fotovoltaico. Vicende così lontane e così diverse che hanno, però, reso evidente come sia una grave carenza per il nostro Paese non essersi dotato della Strategia energetica nazionale a cui si è preferita la strada delle scelte estemporanee (come è stato per il nucleare) o delle stroncature (come è stato per le rinnovabili); scelte che dovevano seguire e non certo anticipare la definizione della strategia in campo energetico del Paese. L'adozione del decreto sulle energie rinnovabili con contenuti del tutto lontani dalle condizioni e dalle osservazioni poste unitariamente ed unanimemente dalle Commissioni parlamentari è non solo incomprensibile e lesiva delle prerogative del Parlamento, ma produce l'effetto di affossare, anziché promuovere, le rinnovabili in controtendenza con le direttive dell'Unione europea e con gli stessi recenti autorevoli auspici del Capo dello Stato. Eppure, solo pochi mesi fa il Governo aveva adottato tre provvedimenti fondamentali: a luglio scorso il Piano di azione nazionale sulle rinnovabili con cui si definivano gli impegni verso il 2020 nei confronti dell'Unione europea; ad agosto il nuovo Conto energia (il terzo) a valere per il triennio 2011-2013 che, tra l'altro, prevedeva una progressiva riduzione degli incentivi, fino al 30 a settembre, infine, dopo ben sette anni di attesa, si approvavano invece le linee guida nazionali. Insomma, finalmente, si dava all'intero settore un quadro normativo, autorizzatorio e di incentivazione, un quadro certo e stabile, capace di tenere insieme gli obiettivi strategici del Paese per lo sviluppo di un settore in forte espansione. Tutto ciò oggi viene nei fatti cancellato, gettando nel panico l'intero segmento industriale delle energie rinnovabili, provocando una vera e propria rivolta, civile ma ferma, cui assistiamo da settimane. Spiace che in questa azione demolitoria si sia speso in particolare il ministro Romani, che, non solo sulla stampa, ma finanche in Commissione industria, si è spinto ad alimentare un clima di ostilità e diffidenza verso il settore diffondendo numeri e dati sui costi degli incentivi che si sono rivelati dei tutto infondati.

Ben altri sono i costi che ancora paghiamo per il *decommissioning* delle vecchie centrali nucleari: 5 euro al mese, da più di venti anni ormai, e ancora per i prossimi dieci. Per non parlare del vero inganno perpetrato ai danni dei consumatori italiani, famiglie e imprese, anche in questo caso da circa venti anni, costituito dal costo in bolletta degli oneri noti come CIP6, costati finora una cifra compresa tra i 40 e i 50 miliardi di euro per sostenere impianti convenzionali o l'industria del petrolio. Altro che costo delle rinnovabili. Ora si tratta di riparare ai gravi danni causati dall'improvvida scelta mossa da furore ideologico, che guarda con fastidio ad una nuova industria dell'energia, e dalle potenti *lobby* che in questa vicenda si sono mosse per orientare la decisione del Governo. Il Governo mantenga l'impegno assunto nelle scorse settimane nei confronti del Paese intero e degli operatori approvare entro i primi giorni del mese di aprile il nuovo Conto energia ed a sanare le contraddizioni più vistose presenti nel provvedimento approvato nei giorni scorsi. Si tratta di ridare linfa ad un settore industriale costituito da circa 2.000 imprese,

stiamo discutendo. Proprio la sciagura che ha colpito la mia terra, le cui immagini hanno impressionato tutta l'Italia, deve farci riflettere sulle innumerevoli difficoltà che oggi sta affrontando quel territorio. In poche ore le Marche hanno visto alcune vie di trasporto strategiche completamente inagibili per lo straripare dei fiumi e il crollo di alcuni ponti. Particolarmente rilevanti anche i danni subiti dalla rete elettrica, che sono stati riconosciuti prontamente dal Governo, che ha immediatamente dichiarato lo stato di calamità naturale per quei territori. Per questo, ora più che mai, è necessario dare un segnale alla popolazione colpita: uno di questi segnali può essere dato proprio dalla salvaguardia di coloro che avevano avviato degli investimenti nel settore del fotovoltaico e che oggi sono impossibilitati a concludere i lavori avviati per le cause di forza maggiore provocate dall'alluvione. In questa direzione si muove l'impegno, che auspico il Governo accolga, a prevedere, per le aree colpite da calamità naturale, così come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 21 marzo 2011, che ha dichiarato lo stato di emergenza, una proroga al 31 dicembre 2011 del termine per la fruizione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010.

Signora Presidente, oggi ci troviamo ad affrontare in Aula un tema molto importante, che è quello delle energie rinnovabili.

audizioni di tutti i soggetti interessati al tema delle energie rinnovabili, si era arrivati alla predisposizione di due pareri, il testo di uno dei quali - voglio ricordarlo - era stato proposto dal Gruppo dell'Italia dei Valori. al parere sul decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 28 del 2009 sulla promozione dell'uso delle energie da fonti rinnovabili, il Gruppo dell'Italia dei Valori, pur evidenziando alcune criticità contenute nel provvedimento, come la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra in area agricola e l'introduzione del meccanismo delle aste al ribasso,

Purtroppo poi il Governo, subito dopo, di fatto ignorando il parere che era stato formulato dalla Commissione competente, e in qualche modo

raggiungimento dell'obiettivo europeo. Tutti sappiamo - ed è stato ripetuto più volte anche in quest'Aula - che l'importanza dello sviluppo delle energie rinnovabili non è soltanto una questione ambientalista, ma è anche una questione di tipo occupazionale, perché sappiamo benissimo che, nell'ipotesi di massimo sviluppo della potenzialità delle energie rinnovabili,

Ho voluto brevemente ricordare quello che è successo sino ad oggi perché è bene, che anche i cittadini sappiano chi è veramente a favore e a sostegno delle energie rinnovabili e chi, come al solito, cioè il Governo Berlusconi, fa degli *spot*, dei proclami e poi, nella sostanza dei fatti, adotta dei provvedimenti che vanno contro le energie rinnovabili. L'Italia dei Valori, come gli altri Gruppi parlamentari, ha presentato oggi per l'Aula una mozione, che la senatrice Carlino ha già illustrato. Vorrei brevemente ripercorrere alcuni punti per parlare poi in particolare del tema delle bioenergie. L'Italia dei Valori, con la mozione che ha presentato, in perfetta continuità e sintonia con il lavoro della Commissione, ha chiesto al Governo di elaborare e fare propria una strategia coerente, stabile ed organica di potenziamento e incentivazione

porre rimedio alle conseguenze, gravi, che si stanno già verificando in questo momento, cioè di evitare che vi sia una sospensione delle linee di credito da parte degli istituti di credito e quindi il blocco degli impianti e la cancellazione di importanti commesse. Abbiamo poi chiesto al Governo di provvedere con urgenza ad una revisione delle strategie energetiche nazionali, alla promozione dell'efficienza e alla riqualificazione energetica nell'edilizia, soprattutto - e abbiamo voluto ribadire questo concetto - abbandonando (dico "abbandonando", non "riflettendo se abbandonare")

almeno per noi dell'Italia dei Valori, è chiaramente una scelta che è maturata solo sull'onda dell'emozionalità della tragedia del Giappone, ma è soprattutto una decisione che pensiamo sia rivolta sia rivolta a depotenziare l'effetto della consultazione referendaria, che - ricordiamo - ci sarà nel mese di giugno. Vengo all'ultimo punto che voglio trattare, ossia il tema delle bioenergie. Nella nostra mozione abbiamo chiesto che si favorisca lo sviluppo delle bioenergie al fine di incrementare la produzione combinata di calore ed elettricità in moderni impianti di piccole dimensioni, secondo un concetto di filiera corta, sottoponendo preventivamente ogni singola iniziativa ad un accurato bilancio energetico comprensivo del trasporto e ovviamente verificando le emissioni di questo tipo di produzione di energia rinnovabile. In ultimo, ma non per importanza, nella nostra mozione si chiede di garantire il mantenimento delle funzionalità essenziali degli ecosistemi interessati. questo passaggio, colleghi, perché l'ho trovato sostanzialmente analogo in tutte le mozioni presentate, ad eccezione di quella presentata dalla Lega. Per evidenziare questa mancanza nella mozione della Lega permettetemi una digressione facendo riferimento alla mia Regione, al Piemonte. Piemonte. In Piemonte è stato sollevato da diversi comitati di cittadini il problema delle bioenergie e in particolare degli impianti di biomasse. nella direzione delle richieste che noi abbiamo evidenziato nella nostra mozione, quindi un'attenzione ai temi che ho ricordato. È evidente che, rispetto a questo sostegno alle richieste dei cittadini, in Piemonte tutte le forze politiche, compresa la Lega, hanno sostenuto la richiesta di moratoria da parte dei cittadini piemontesi. Peccato che, ancora una volta, la Lega dimostri che sui territori dice una cosa, poi viene a Roma e ne dice un'altra. Credo che la mancanza di un'indicazione sulle bioenergie nella mozione della Lega sia il comportamento diverso sui territori e qui a Roma.

la discussione che stiamo svolgendo abbia molto a che fare con i due fatti che da giorni monopolizzano l'attenzione dell'opinione pubblica nel mondo: da una parte, i sommovimenti politici nel Nord Africa e, dall'altra, la tragedia giapponese. Da una parte, le vicende complicate che stanno attraversando il mondo arabo ripropongono, tra gli altri temi, anche il punto dell'insicurezza geopolitica di sistemi energetici come il nostro, largamente dipendenti da fonti fossili importate; dall'altra parte, la catastrofe di Fukushima, di cui ancora oggi non sappiamo quali saranno le conseguenze (ma sappiamo che saranno in ogni caso drammatiche), richiama un altro nodo delicato, ossia l'insicurezza tecnologica dei sistemi energetici che fanno largo ricorso alla produzione elettronucleare. Accanto ai problemi dell'impatto ambientale e climatico dell'energia prodotta bruciando petrolio ed altri combustibili fossili, queste due grandi emergenze planetarie ribadiscono l'urgenza di una transizione energetica orientata in due principali direzioni: migliorare l'efficienza degli usi dell'energia e diffondere l'uso delle fonti energetiche rinnovabili. Si tratta in entrambi i casi di direzioni tecnologicamente sicure e ambientalmente sostenibili, direzioni indispensabili per affermare la sovranità energetica di Paesi come l'Italia, dove sole, vento, acqua, geotermia sono le sole fonti energetiche di larga disponibilità. Il punto, se si parla di fonti rinnovabili, è quanto costi alla collettività promuovere l'uso delle energie pulite, a cominciare dal solare fotovoltaico che è la più promettente, ma anche quella che oggi richiede il sostegno più rilevante. Su questo, circolano spesso dati improbabili, come ricordava il senatore Ferrante illustrando la nostra mozione. In base ai dati ufficiali del GSE (che hanno il loro peso), nel 2010 il peso delle rinnovabili sulla componente A3 delle bollette elettriche pagate dagli italiani è stata di 2.700 milioni; di questi, 826 milioni riguardano il fotovoltaico: 826 milioni sono una cifra molto inferiore a quanto gli utenti hanno pagato per sostenere le fonti cosiddette assimilate, come l'energia dai rifiuti, ed incomparabilmente meno di quanto costa agli italiani sostenere molti altri comparti produttivi non altrettanto strategici. D'altra parte, è proprio grazie agli incentivi se il mercato del fotovoltaico, diffondendosi, può progressivamente abbassare i suoi costi. Se oggi in Germania gli incentivi sono più bassi che in Italia, come da più parti viene ricordato, è perché per anni il settore in Germania è stato fortemente sostenuto, facendo di quel Paese il leader mondiale, sia nei consumi che nella produzione dei pannelli. Se come ha dichiarato ieri il commissario europeo che si occupa dei cambiamenti climatici, l'eolico *off shore* già oggi è meno costoso del nucleare, la ragione è la stessa: soltanto gli investimenti, la nascita di una filiera industriale, produce rapidamente un abbassamento dei costi. L'Europa sta puntando molto sulle rinnovabili, con obiettivi decisamente più ambiziosi di quelli, di base, fissati dall'Unione europea al 2020: lo fa non perché è più buona degli altri, ma perché sa che questa è, in primo luogo, una grande sfida per l'innovazione tecnologica, per la competitività dei nostri sistemi economici.

a crescere in questi anni di crisi, con migliaia di imprese che danno lavoro a oltre 100.000 persone. Per questo ritengo che sia nell'interesse di tutti rimediare rapidamente a questo grave con norme che devono certamente dimostrarsi equilibrate, che tengano conto dei progressi della tecnologia e del conseguente abbassamento del costo delle rinnovabili, ma che non ci facciano rinunciare a una prospettiva che considero letteralmente irrinunciabile, ossia fare dell'Italia uno dei grandi Paesi delle energie pulite nel mondo. Questo è un indiscutibile e prioritario interesse strategico del nostro Paese e mi auguro che il Governo, ascoltando e prendendo lezione ed insegnamento dai contenuti delle mozioni presentate oggi, nel momento in cui nei prossimi giorni dovrà riparare all'errore commesso, tenga conto di questa banale verità.

a prevedere che, per entrata in esercizio, si intenda il «fine lavori dell'impianto e delle opere di connessione alla rete», così come asseverato da un tecnico abilitato; per gli impianti completati dopo tale data a definire un periodo transitorio con incentivi decrescenti; Questa è la riformulazione proposta, rispetto alla quale chiediamo il parere del Governo.

il costo del kilowattora è straordinariamente importante per la nostra economia. La voce A3, un prelievo obbligatorio sulla bolletta elettrica, incide ormai intorno al 10 per cento complessivo del costo del kilowattora, nel nostro Paese è già elevato. Bisogna avere molta attenzione a non incrementare ulteriormente questo fondamentale costo per la nostra economia, che è un'economia che deve vivere di esportazioni. il decreto ministeriale 6 agosto 2010, che prevede l'incentivazione del fotovoltaico per gli anni 2011, 2012 e 2013, 3, comma 2, afferma che la potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti, di cui al titolo II del decreto, tale soglia. Il precedente conto energia, che è un decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, stabiliva che la potenza massima cumulata

non attraverso un prelievo fiscale come in questo caso, ma comunque attraverso un prelievo obbligatorio, debba essere indicata complessivamente la somma che viene ad essere prelevata.

Presidente, riteniamo molto grave la situazione che si è determinata per il fatto che, su un tema di tale rilevanza, sul quale vi è l'attenzione di tutto il Paese,

Dopodiché, Presidente, siccome ci interessa conseguire un risultato serio, nell'interesse del mondo delle energie rinnovabili, non saremo noi a determinare il fallimento dell'operazione. Abbiamo a cuore, infatti, le sorti di questo settore dell'economia

la votazione con sistema elettronico, è verosimile che la parte che il Ministro ha ritenuto di espungere dalla nostra mozione, ossia quella che prevede un ripensamento e quindi un abbandono della strategia nucleare da parte del Governo, non

sia per la politica energetica del Paese sia per quanto riguarda legittimi interessi che sono in campo da più parti. Dobbiamo una risposta a cittadini, imprenditori e lavoratori,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro, la giornata di oggi affronta un tema particolarmente condiviso da tutte le forze politiche, che riprende con serietà un argomento che negli ultimi tempi sembrava caduto in prescrizione, ossia il problema della politica energetica nel nostro Paese. Oggi noi ci preoccupiamo di attirare l'attenzione sulla necessità di incentivare la politica delle energie rinnovabili

degli ultimi giorni con cui si era drasticamente intervenuti tagliando gli incentivi per la produzione delle energie rinnovabili, così determinando un gravissimo danno.

Il colpo di mano del Governo, con l'azzeramento degli incentivi, avrebbe determinato un effetto immediato per il lavoro programmato e finanziato, che riguarda oltre 15.000 addetti: improvvisamente, a contratto in corso, si chiudevano i rubinetti, mettendo in crisi un settore. Ma questo è uno degli aspetti, il più immediato. Il problema più importante è invece che oggi, leggendo tutte le mozioni, prende vigore la politica delle energie rinnovabili, che nel nostro Paese ha subito, purtroppo, fasi di attenzione altalenanti. Ho ancora memoria di quando, nel 2005, con un colpo di mano, un decreto del presidente del Consiglio Berlusconi licenziava il presidente dell'ENEA, che portava avanti il programma delle energie rinnovabili, in modo particolare del solare termodinamico. Lo licenziava

Poi, il nostro progetto, frutto del genio italiano, è stato ripreso dalla Germania con il programma Desertec, che prevede un investimento di 400 miliardi di euro per un grande impianto da realizzarsi e che produrrà energia solare nella misura del 15 per cento del fabbisogno europeo. Con le nostre invenzioni gli altri realizzano l'energia rinnovabile, abbandonando quel programma, abbiamo perso anni, perché vi è stata una timida ripresa nel 2008, quando venne richiamato il professor Rubbia come consulente si arrivò ai decreti ministeriali, il 28 marzo 2008, con cui venivano individuate le quattro Regioni con i progetti sperimentali del solare termodinamico (Sardegna, Calabria, Lazio e Puglia).

sulle energie rinnovabili, impegnando il proprio Paese ad assicurarsi un approvvigionamento nella misura pari all'80 per cento del fabbisogno attraverso le rinnovabili. Noi invece siamo l'unico Paese

assistere alla presa in giro di una moratoria di un anno, fatta soltanto, come il ministro Prestigiacomo ha candidamente ammesso in un fuori campo captato,

Questo è un inganno al popolo italiano ed una presa in giro. È un discorso cinico, ma gli italiani, il 12 giugno, spazzeranno via la vostra prepotenza prepotenza e arroganza votando sì al *referendum* per l'abolizione del nucleare e contro i pasticcioni, imbroglioni e coltivatori di *business*.

Presidente, avendo illustrato ampiamente la mozione mi limiterò ad una brevissima dichiarazione di voto. Ritengo che il Governo debba procedere ad eliminare appunto anche quegli scarti

una migliore definizione degli incentivi che saranno caricati attraverso il nuovo conto energia sulle energie rinnovabili, ritenendo che una politica coerente non possa prescindere non solo dal sostenere le energie rinnovabili, ma anche da una concezione ampia, moderna che usi le nuove tecnologie in maniera sicura e sostenga la ricerca scientifica e tecnologica in questo campo. Quindi, siamo anche, e soprattutto, per il sostegno alle innovazioni di progetto e per il sostegno anche alla ricerca in questo settore. Non limitiamoci soltanto a questo discorso *tout court*, necessario e doveroso rispetto alle energie rinnovabili ed alla legge che dovrà regolamentare gli incentivi che dovranno essere parte del nuovo decreto, ma guardiamo anche oltre. E guardando oltre, dobbiamo vedere come il nostro Paese debba assolutamente affrancarsi dalla dipendenza energetica affrontando la questione dell'energia ad ampio raggio, senza paure o condizionamenti emotivi, ma con la razionalità e la prudenza necessarie perché effettivamente si possa migliorare la qualità della vita, dare una sicurezza allo sviluppo incentivandolo attraverso un minore costo della stessa energia ed utilizzando tutte le fonti più appropriate

le mozioni che abbiamo discusso oggi sono state presentate per porre un quadro di riferimento al Governo affinché vengano corretti degli errori che evidentemente sono stati commessi nel recepimento della direttiva comunitaria sulle rinnovabili. Credo che la discussione di oggi abbia messo in evidenza una convergenza sostanziale da parte dei Gruppi parlamentari su un tema che ha una rilevanza strategica e che nessun Gruppo ha sottaciuto. C'è quindi da augurarsi che la discussione di oggi e il contenuto delle mozioni possano rappresentare la premessa unitaria per la definizione di una strategia energetica matura, consapevole, libera da condizionamenti ideologici e tesa a determinare le condizioni perché, combinando la tutela ambientale con lo sviluppo industriale, si possa ricollocare il nostro Paese in una posizione rilevante nello scenario europeo. È importante rilevare come una strategia energetica non solo debba fare riferimento al *mix* delle fonti e debba valorizzare le componenti tecnologiche connesse alle politiche di generazione dalle rinnovabili, ma debba anche mettere in campo tutte le azioni positive tese a garantire il risparmio e l'efficienza e, da questo punto di vista, porre all'attenzione del Paese il tema della microgenerazione distribuita, valorizzando le acquisizioni ingegneristiche e tecnico-scientifiche che oggi ci consentono di puntare alla cogenerazione e alla trigenerazione combinando insieme queste modalità con il fotovoltaico e con il solare termodinamico. Tutto ciò costituisce la premessa fondamentale perché si possa guardare al sistema di trasmissione e di connessione del nostro Paese con il il resto dell'Europa in termini di efficienza, utilizzando le reti intelligenti che si complementano fortemente con la produzione distribuita da fonti rinnovabili. C'è da augurarsi quindi che gli impegni assunti in sede comunitaria possano rappresentare una straordinaria opportunità di crescita e di sviluppo industriale per il nostro Paese. Le mozioni presentate collocano la riflessione del Parlamento su questo livello; per questo noi esprimeremo un voto favorevole su tutte le mozioni presentate.

presentata dal senatore Molinari sono state accolte; quindi tutto sommato ci dichiariamo soddisfatti. Fondamentalmente, a noi interessava segnalare come la vicenda delle energie rinnovabili resti, nel quadro delle esigenze energetiche del nostro Paese, la via principale e la pista da perseguire con volontà, con tenacia e con coerenza da parte di tutto

liquidare il nucleare in quattro righe sia oggettivamente eccessivo. Noi pensiamo che il tema e la questione, che occupano gli spazi delle discussioni ormai non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei cittadini (per le note vicende), meritino un approfondimento diverso

mare*. Signora Presidente, io non ho chiesto la votazione per parti separate. Ho dato un parere favorevole, a condizione che venissero espunti i due punti che ho precisato. Questa richiesta non è stata accolta; di conseguenza il parere si intende contrario.

Grazie, signor Presidente. consolidando un orientamento della giurisprudenza, ha condannato la CONSOB del signor Cardia per omessa vigilanza. La Cassazione ha affermato che la CONSOB deve svolgere la sua attività sia nel rispetto delle norme speciali che la riguardano, sia nell'osservanza del principio ordinario del *neminem da collegare alle misure costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione. In tale prospettiva, la Commissione è soggetta al rispetto dell'articolo 2043 del codice civile sulla produzione del danno ingiusto e sul conseguente risarcimento. In questa Aula ho spesso denunciato i comportamenti di una gestione sciagurata della CONSOB di Cardia, di Maccarone e di Salvini; era capo dell'ufficio legale, e che invece di vigilare preventivamente sui danni che si andavano a produrre e sulle truffe del risparmio tradito,

dal Governo a rispondere per omessa vigilanza? Farà un'azione di responsabilità affinché quei danni che sono stati inferti vengano pagati da loro,

e per le contiguità di Cardia, della CONSOB e della Banca d'Italia. Signora Presidente, una semplice comunicazione, che avrei potuto fare ieri sera, ma non è stato possibile. Come concordato nella riunione dei Capigruppo, le inoltro l'indicazione dei disegni di legge che il Gruppo UDC, SVP, Autonomie, Repubblicani intende fare propri, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, chiedendone l'inserimento nel calendario dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, terzo periodo, del Regolamento: n. 1287 («Modifica alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale); n. 2583 («Trasferimento del punto franco istituito nella zona falcata del porto di Messina con legge 15 marzo 1951, n. 191»); n. 1113 («Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»); n. 2416 («Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti politici»).

Volevo intervenire su una questione seria, visto che era presente anche un esponente del Governo. Poco tempo fa

rispetto ad un allargamento che comporta spese e maggiori costi della politica. Si sono aggiunti altri tre assessori per fare un piacere politico ad un sindaco perché non è riuscito a comporre una maggioranza organica con solo 15 assessori: mi chiedo se non sia il caso di approfondire questa vicenda con un dibattito,

riguarda le fermate dell'Eurostar nella stazione di Spoleto, che da più di un anno sono state escluse dalla linea Orte-Falconara e i pendolari devono aspettare più di un'ora da Terni a Spoleto per poter raggiungere la propria casa. È una situazione veramente grave.